L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

ha comunicato che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato, ha verificato, nella seduta del 25 settembre 2018, la sussistenza dei titoli indicati nel decreto presidenziale, in data 19 gennaio 2018, recante la nomina a senatrice a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, della dottoressa Liliana Segre, per avere illustrato la patria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

Restano confermati per le sedute di questa settimana l'esame dei disegni legge di rendiconto e assestamento - che saranno discussi oggi pomeriggio - e il sindacato ispettivo.

il Ministro degli affari esteri renderà l'informativa sugli sviluppi della situazione in Libia. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la ratifica Italia-Abu Dhabi su estradizione e assistenza giudiziaria nonché, ove conclusi dalla Commissione, i disegni di legge sullo sviluppo delle isole minori. Nella settimana dal 9 all'11 ottobre saranno discussi la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 nonché, ove conclusi dalle Commissioni, l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, i disegni di legge sulla rete nazionale dei registri dei tumori e sul voto di scambio politico-mafioso. Martedì 16 ottobre, alle ore 9,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre. Il calendario della settimana prevede inoltre la discussione, ove conclusi dalle Commissioni, dei disegni legge sull'educazione civica nelle scuole, sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e sulla legittima difesa. Tutti i disegni di legge di iniziativa parlamentare previsti dal calendario provengono dalla sede redigente. Peraltro - dopo la conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo i disegni di legge concernenti la legittima difesa sono stati rimessi alla sede referente per iniziativa di un quinto dei senatori della Commissione giustizia. Su tale questione sarà riconvocata la Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, in raccordo con l'articolo 74, comma 3, del Regolamento, tenuto conto del fatto che uno dei provvedimenti è di iniziativa popolare. Il calendario dei lavori prevede, per ciascuna settimana, sedute di sindacato ispettivo e ogni giovedì, alle ore 15, il *question time*. Il calendario potrà, infine, essere integrato con la votazione di nove componenti effettivi e nove supplenti della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Ai fini di una più agevole programmazione dei lavori delle Commissioni, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che le sedute saranno sospese, in linea di massima, tra le ore 13,30 e le ore 16,30, fermi restando gli orari del *question time*.

ha correttamente riferito che il calendario è stato approvato a maggioranza, ho quindi una proposta da fare all'Assemblea di modifica del calendario che lei ha ricordato a tutti noi. A norma dell'articolo 55, comma 3, le chiedo di anticipare il provvedimento che istituisce la Commissione d'inchiesta sul femminicidio alla settimana prossima, potrebbe essere lo stesso 2 ottobre subito dopo l'informativa sulla Libia o, in alternativa, il giorno successivo. Ho colto la disponibilità dei colleghi Capigruppo, in buona fede, di dare seguito positivamente a questa istituzione. C'è un accordo che riguarda, mi sembra, tutti i Gruppi politici,

che sia un tentativo latente di svuotamento dell'attività parlamentare, ma di questo non parliamo oggi, ne parleremo in un'altra occasione. Oggi mi voglio limitare a chiedere all'Assemblea questa modifica su un tema così rilevante, come, ahimè, la cronaca

finestra"). Prima di passare alla votazione della proposta del senatore Marcucci, è facoltà per chi lo desidera di intervenire uno per Gruppo.

con tutto il rispetto, la posizione del presidente del MoVimento 5 Stelle. Sappiamo benissimo che le altre Commissioni sono state

proprio dal Senato durante la scorsa legislatura, che ha visto partecipi tutte le forze politiche in maniera trasversale, una Commissione che anche questa volta nasce con trasversalità e con obiettivi con obiettivi condivisi da tutti. Vorrei comprendere il motivo della discussione, perché si tratta di obiettivi compresi, condivisi da tutti e già affrontati da chi ha

calendarizzato per la settimana successiva e noi abbiamo fatto uno sforzo, parlando direttamente con il Presidente della Commissione, per arrivare al 9 ottobre. Cosa cambia esaminarlo una settimana dopo? È solo per un motivo tecnico, per dare la possibilità che ci sia la discussione,

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vi relaziono sul «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2017». Com'è noto, il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto generale dello Stato, è articolato per missioni e programmi. È costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. In attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, al «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato» è allegata, per ciascuna Amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, la nota espone le risultanze della gestione per ciascun programma di spesa, in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione. Più precisamente, la nota integrativa, con riferimento alle azioni sottostanti a ciascun programma, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. Essa contiene, inoltre, l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi della spesa, misurato attraverso appositi indicatori che potrebbero costituire la base per una compiuta analisi dell'attuazione delle politiche pubbliche da parte delle amministrazioni preposte. Il rendiconto generale dello Stato è inoltre corredato dal rendiconto economico al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato e di una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato (il cosiddetto ecorendiconto dello Stato). Venendo al contenuto del disegno di legge di rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, si segnala che, nel suo insieme, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2017 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive contenute nell'assestamento 2017. A raffronto con l'esercizio precedente, invece, i dati di consuntivo evidenziano un peggioramento sia del saldo netto da finanziare, che del ricorso al mercato. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2017 un valore negativo per 29,1 miliardi cento del PIL), con un peggioramento di circa 18 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2016 (-11,1 miliardi), dovuto al sensibile aumento delle spese finali e, in particolare, di quelle in conto capitale (oltre 20 miliardi), nettamente superiore rispetto all'incremento delle entrate finali. Tale saldo è tuttavia risultato migliore delle previsioni definitive per oltre 24,6 miliardi di euro. Si registra, invece, un miglioramento del risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti), il quale passa dai 27,8 miliardi di euro registrati nel 2016 a un valore di 31,6 miliardi cento del PIL), con un miglioramento di circa 3,8 miliardi rispetto al 2016. Tale situazione si è determinata a causa di una diminuzione delle spese correnti (-0,7 miliardi) rispetto al complesso delle entrate tributarie ed extratributarie (+3 miliardi). Il miglioramento è marcato anche con riferimento alle previsioni definitive (circa 6,9 miliardi). Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2017 a 271,2 miliardi (con un'incidenza sul PIL del 15,8 per cento), evidenziando un aumento rispetto al 2016 (+207,1 miliardi di euro), dopo una tendenza alla diminuzione registrata negli ultimi anni a 260,4 miliardi nel 2014 e a 257,1 miliardi nel 2015). Il valore del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato registrati nel 2017 si mantiene comunque al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bilancio per il 2017

e a -310.682 milioni per il ricorso al mercato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a seguito degli effetti peggiorativi dovuti agli interventi di sostegno del sistema bancario). Dal lato delle entrate finali, l'incremento degli accertamenti (pari a 1,7 miliardi di euro) è ascrivibile per la maggior parte alle entrate tributarie e in misura minore a quelle extratributarie. Guardando alle entrate complessive, l'entità degli accertamenti (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata nel 2017 pari a 864,6 miliardi di euro, con un forte incremento rispetto al 2016 (+2,2 per cento, pari a +18,6 miliardi), che trae origine soprattutto dalla dinamica degli accertamenti delle entrate del titolo IV (Accensione prestiti). Su tale voce si registra, infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'aumento di 20 miliardi di euro, derivante dall'attuazione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio». L'incidenza sul PIL è pari al 50,4 per cento per gli accertamenti complessivi, in linea con quanto fatto registrare lo scorso anno (50,6 per cento del PIL nel 2016). Dal lato della spesa, si rileva un aumento degli impegni finali di spesa nel 2017 (pari a 612,1 miliardi di euro) per un ammontare di 19,6 miliardi: tale tale risultato è frutto di una lieve contrazione delle spese correnti (-0,7 miliardi) e di un notevole incremento della spesa in conto capitale (+20,4 miliardi) rispetto al 2016, da attribuire prevalentemente alla categoria «Acquisizione di attività finanziarie», per effetto dell'attuazione del citato decreto-legge n. 237 del 2016, che consolida il *trend* positivo iniziato lo scorso anno dopo il forte calo registrato tra il 2014 e il 2015. Venendo alla gestione dei residui, si rammenta previamente che l'andamento dei residui passivi registrato per il 2017 risente del nuovo regime contabile dei residui passivi introdotto dal decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha determinato un aumento del termine di conservazione in bilancio dei residui propri, portandolo da due a tre anni per i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4 del titolo I) e per le spese in conto capitale (titolo In base ai dati forniti nella relazione al rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti indicava al 1° gennaio 2017 residui attivi presunti per un valore di 212.238 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 134.423 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti, con un'eccedenza attiva pari a 77.815 milioni di euro; nel 2016 l'eccedenza attiva era di valore superiore, pari a 95.229 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio 2017 l'entità dei residui si è andata modificando a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, che ha fatto registrare variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate, per 62.209 milioni di euro, sia dal lato delle uscite, con una diminuzione di 17.590 milioni di euro. Pertanto, rispetto allo *stock* iniziale di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti

A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza dell'esercizio 2017, circa 88.263 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2017 pari a 204.076 milioni Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, su 234.423 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2017 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 116.833 milioni, di cui di cui 49.089 milioni pagati e 67.744 milioni ancora da pagare. Tali residui pregressi, unitamente ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2017, 2017, risultati pari a 70.161 milioni di euro, determinano un totale complessivo di residui passivi al 31 dicembre 2017 di 137.905 milioni. Scorporando la quota di residui passivi relativi al titolo III, concernenti il rimborso delle passività finanziarie, pari a 475 milioni, i residui passivi delle spese finali ammontano a 137.430 milioni. In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2017, espone residui attivi per 204.076 milioni di euro e residui passivi per 137.905 milioni di cui 475 milioni relativi al titolo III, concernenti il rimborso delle passività finanziarie. Per quanto riguarda il conto generale del patrimonio, il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato quale risulta alla chiusura dell'esercizio, dai risultati 2017 emerge un'eccedenza passiva di circa 1.875 miliardi, con un peggioramento di oltre 77,4 miliardi Si tratta di un risultato che continua il *trend* degli ultimi tre anni, considerato che nel 2016, sul 2015, il peggioramento è stato di poco inferiore ai 40 miliardi e nel 2015, sul 2014, pari a meno 66,8 miliardi Il totale delle attività ammonta circa 947,8 miliardi, di cui 736,5 miliardi di attività finanziarie, in netta diminuzione rispetto a 2016, e 307 miliardi di attività non finanziarie.

Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2016, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 38,2 miliardi di euro. Concludo, tenendo conto delle criticità negative soprattutto evidenziate alla voce «Conto generale del patrimonio», invitando a prestare una maggiore attenzione alla scelta degli obiettivi adottati dalle amministrazioni, collegandoli più strettamente al raggiungimento in tempi brevi dei risultati positivi, misurabili attraverso una rapida ripresa economica sostenibile per la Nazione, garantendo il risanamento dei nostri conti pubblici.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, la 5ª Commissione ha esaminato in sede referente il disegno di legge recante le disposizioni per l'assestamento del bilancio, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato per missioni e programmi, costituenti le unità di voto, ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo definito dalla legge di contabilità, così come modificata e integrata dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016. Tali modificazioni, però, non hanno comunque interessato la natura del provvedimento in esame, che resta una legge formale, costituita dalla sezione II della legge di bilancio. In sede di assestamento possono essere modificati gli stanziamenti di spese predeterminate per legge (la cosiddetta flessibilità di bilancio), fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. I margini di flessibilità in sede di assestamento sono stati recentemente ampliati a seguito delle modifiche, introdotte prima col decreto legislativo n. 90 del 2016 e poi dall'articolo 5 della legge n. 163, sempre del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica. Tali modifiche consentono di proporre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra unità di voto diverse, laddove la flessibilità era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione. La legge sopra citata, la n. 163 del 2016, ha inoltre previsto, a partire dal 2017, che anche il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, nella quale si dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Documento di economia e finanza. Sul punto, giova segnalare che la relazione tecnica relativa all'odierno disegno di legge non necessita dell'aggiornamento previsto, ai sensi del comma 4-*septies*, dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, in quanto gli emendamenti approvati non mutano il quadro contabile già rappresentato al momento della presentazione del disegno di legge in esame. Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2018, indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle amministrazioni autonome. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione in termini di competenza e di cassa delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento e per ciascuna unità di voto si indicano inoltre le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto. L'articolo 2, comma 1, innalza di 2 miliardi di euro per il 2018, portandolo da 18 miliardi di euro a 20 miliardi Il Governo, specificamente interrogato, ha chiarito che l'incremento del limite degli impegni di SACE di durata superiore a ventiquattro mesi, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato, non ha effetti su fabbisogno e indebitamento netto, in quanto, trattandosi di garanzie cosiddette non standardizzate, la contabilizzazione delle operazioni a peggioramento dei predetti saldi è solo eventuale, nel caso in cui le garanzie fossero effettivamente escusse: pertanto non si sconta alcun effetto sui predetti saldi. Il comma 2 novella invece il comma 5 dell'articolo 3 della legge di bilancio, recante la quantificazione degli importi dei Fondi inseriti nel programma Fondi di riserva e speciali,

L'articolo 3 novella l'articolo 9, comma 3, della legge di bilancio, al fine di introdurre l'esatta denominazione del programma, riconducibile alla missione Ordine pubblico e sicurezza, all'interno del quale sono allocate le somme attribuite al fondo dedicato alla ridotazione di risorse per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, in particolare il capitolo 2676. La denominazione qui proposta è «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», in luogo della denominazione «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», attualmente riportato dal testo della legge di bilancio. L'articolo 4 reca invece due novelle all'articolo 18 della legge di bilancio, contenente disposizioni diverse aventi per lo più carattere gestionale. Per quanto riguarda i risultati finanziari determinati dal disegno di legge di assestamento per il 2018, si segnala che la relazione evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio che si attesta a un valore di meno 43,8 miliardi, rispetto a una previsione iniziale di meno 45 miliardi. Il miglioramento di circa 1,2 miliardi di euro del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali è dovuto essenzialmente all'effetto positivo, per 2,45 miliardi di euro, derivante dalle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, compensato per meno 1,2 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo. Il miglioramento del saldo netto da finanziare, che si determina nelle previsioni assestate in termini di competenza rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto a un decremento delle spese finali per 2,2 miliardi di euro. Infatti queste passano da 624.554 a 622.332 milioni di euro, parzialmente compensate da una riduzione delle entrate finali di quasi un miliardo di euro. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 1,2 miliardi in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali (più 1,3 miliardi). Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico registra un miglioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 3,7 miliardi. Con riguardo alle proposte di variazione formulate con il disegno di legge di assestamento, le stesse vanno distinte tra quelle concernenti le entrate e quelle relative alle spese. Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 1.120 milioni di euro. Per quanto concerne le spese finali, che - come detto - diminuiscono complessivamente di 2,2 miliardi, le variazioni proposte dal provvedimento determinano una riduzione di 3.570 milioni di euro. Tale riduzione interessa esclusivamente le spese correnti, che diminuiscono di 4.210 milioni di euro, nel cui ambito si registra una significativa proposta di diminuzione di quelle per interessi (meno 3.171 milioni), legata per 2.271 milioni alle minori esigenze relative al pagamento di interessi sui titoli pubblici, nonché, per 900 milioni, alle minori esigenze per gli interessi sui conti correnti di tesoreria. La spesa in conto capitale registra invece un incremento di 640 milioni. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati approvati tre soli emendamenti al disegno di legge di assestamento 2018. Si tratta di un emendamento che ha destinato 500.000 euro al programma 12.2 del MEF di sostegno allo sviluppo sostenibile, di un altro emendamento del Governo finalizzato a rifinanziare per 10 milioni di euro il settore dello spettacolo dal vivo e della sostituzione della denominazione della tabella n. 12 con la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo« invece di «Ministero per i beni e le attività culturali». Alla luce delle superiori considerazioni, la 5a Commissione ha licenziato con esito favorevole il disegno di legge in discussione. Si invita pertanto l'Assemblea a voler procedere alla sua approvazione.

il rendiconto e il conto economico dello Stato permettono di verificare gli impegni assunti, i risultati rispetto alle previsioni iniziali il rispetto dei vincoli europei sull'indebitamento netto e il debito pubblico. Dai dati che anche i relatori hanno evidenziato poco fa, emergono chiaramente alcuni numeri e alcuni dati precisi e incontrovertibili. Il PIL, cioè il reddito e la ricchezza complessiva del Paese, ha registrato una crescita del 2,1 per cento rispetto al 2016 e il PIL reale dell'1,5. È dal 2014 che il nostro Paese non è più in recessione, e la crescita ha registrato punti di avanzamento in ognuno di questi anni, toccando nel 2017 il suo apice dopo la crisi. Questa crescita sostenuta anche nello scorso anno ha comportato un netto incremento delle entrate correnti rispetto al 2016. Se guardiamo i saldi di finanza pubblica, l'indebitamento netto, il *deficit* ha raggiunto quota 39.691 miliardi; al netto delle risorse che sono state destinate alla copertura dei problemi del sistema bancario, l'indebitamento netto nel 2017 è stato pari a 33.184 miliardi, cioè all'1,9 per cento del PIL, quindi l'indebitamento netto migliora sia in termini assoluti nel 2016 il valore era di 41,638 miliardi - sia in termini relativi, passando dal 2,5 per cento del PIL all'1,9 per cento. Questo importante risultato è stato raggiunto con un miglioramento di 1,1 miliardi del saldo primario e con una riduzione di 0,87 miliardi della spesa per interessi, ovviamente ottenuta grazie alla credibilità internazionale del nostro Paese che ha permesso sui mercati finanziari di ottenere tassi più bassi e uno *spread* contenuto. Il miglioramento del saldo è determinato principalmente da un incremento delle entrate per 12,1 miliardi, pari all'1,5 incremento più che compensativo della crescita della spesa, che è stata pari a 10 miliardi, che ha corrisposto a un incremento dell'1,2 per cento Una spesa che, però, è cresciuta principalmente nella sua componente di investimenti per 7 miliardi e di circa 3 miliardi per la parte di spesa corrente, quindi portando ulteriore beneficio al ciclo economico del Paese. A fronte dell'incremento delle entrate, come abbiamo detto, però, la pressione fiscale si è ridotta di 0,2 punti percentuali, come, del resto, viene messo in evidenza nella relazione stessa e nel *dossier* a pagina 13: è passata dal 42,7 per cento del PIL nel 2016 al 42,5 per cento nel 2017. Se dovessimo nettare questi importi da quello che è il cosiddetto bonus di 80 euro, la pressione fiscale nel 2017 Il debito pubblico nel 2017 è cresciuto a quota 2.263,056 milioni di euro, con un incremento di 43.150 milioni rispetto all'anno precedente, ma il dato che rileva ai fini del rispetto dei vincoli europei è la sua incidenza sul PIL, che è diminuita di 0,2 punti percentuali, passando dal 132 per cento del 2016 al 131,8 cento del 2017. Si tratta del secondo anno consecutivo di riduzione del rapporto debito-PIL rispetto alla veloce crescita conseguente la crisi economica e la drastica diminuzione del PIL che si è registrata negli anni dal 2008 al 2013. Per quanto concerne la gestione di competenza, nel 2017 essa ha fatto registrare un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive. Nel complesso, quindi, sono aumentate le entrate fiscali,

rimanendo però entro i parametri europei che l'Italia si è impegnata a rispettare. Al netto di questi dati, qualche considerazione politica, ovviamente, va fatta. In questi giorni il Vice *Premier* ha dichiarato che il PD ha distrutto il Paese: i dati positivi che anche i relatori hanno messo in evidenza ci fanno dire che forse la realtà è piuttosto diversa da quella che viene rappresentata con dichiarazioni clamorose. Il PD ha raccolto una condizione di grandissima difficoltà del Paese nella peggiore crisi economica che l'Italia ha vissuto dal Dopoguerra: ha saputo accompagnarlo tirandolo fuori dalla crisi e portando a casa i risultati che oggi, nel rendiconto 2017, vengono ben fotografati. Io ho fatto l'amministratore locale per dieci anni e anch'io mi sono scontrato ogni anno, nell'elaborazione del bilancio, con i vincoli della finanza pubblica, peraltro decisi dal Parlamento;

Un bilancio è fatto di programmi, di missioni, di capitoli e un politico è chiamato a svolgere la sua funzione fino in fondo, che è quella di scegliere cosa poter fare con le risorse limitate che sono a disposizione. Quando sento dire che si vuole aumentare il *deficit* quest'anno per poter rispondere alle tante promesse elettorali, per poi rientrare dal *deficit* e dal debito nei due anni seguenti, mi chiedo se si abbia piena coscienza della differenza tra spesa corrente e spesa per investimenti. Fare *deficit* per finanziare una misura di spesa corrente significa doverla garantire anche negli anni a seguire. Diverso è fare *deficit* per fare investimento, che peraltro produce ulteriore ricchezza nel Paese. Sarebbe stato forse utile che il contratto di Governo, che la maggioranza parlamentare ha siglato, fosse stato fatto dopo l'approvazione del consuntivo, che fotografa la condizione precisa

invitando, anzi sfidando la maggioranza a dimostrare con le proprie capacità, con le proprie competenze, con le proprie scelte politiche quanto sarà in grado nel rispetto dei limiti che la finanza pubblica e che i parametri europei ci impongono. Lo vedremo sicuramente negli anni a venire e verrà fotografato nei consuntivi dei prossimi anni.

cercherò di rendere meno arida questa discussione generale dandovi alcuni dati di sintesi del nostro rendiconto 2017 e dell'assestamento 2018. Una premessa al collega che mi ha appena preceduto: qualcosa deve non aver funzionato, nel senso che, se, come egli tutti "oro" i numeri che in questa sede oggi rappresentiamo, non si capisce perché i cittadini italiani, nel corso delle ultime elezioni politiche, abbiano scelto una maggioranza completamente diversa.

cento del PIL del nostro Paese. Già questi due dati danno la stura ad alcune considerazioni generali. È vero, l'indebitamente netto del nostro Paese diminuisce nel quadriennio 2014-2017, passando dal 3 per cento L'ultimo dato importante è la drastica riduzione degli oneri sul debito, scesi a 65 miliardi e mezzo (erano 74 nel 2014): sono i minori interessi passivi che paghiamo per effetto della politica monetaria della Banca centrale effetto della politica monetaria della Banca centrale europea. Questi sono i dati di sintesi. Come Gruppo Forza Italia rileviamo, però, alcune criticità, sia in relazione al rendiconto, sia in relazione all'assestamento. Questo Governo, che è stato definito «del cambiamento», non ha, a oggi, adottato alcun provvedimento che aiuti realmente l'economia italiana a rialzarsi. Gli scenari macroeconomici sono in rapido peggioramento: chi sta male, sta sempre peggio, chi sta bene sta sempre meglio. Pertanto servono interventi urgenti, di programmazione economica precisa, con una chiara e netta inversione di tendenza che a oggi non notiamo. Serve che il Governo annunci una strategia credibile per ridare fiducia agli investitori, per lo più stranieri, e speranza agli italiani. Ad oggi solo annunci roboanti, più per i titoli dei giornali e per i *social network*, con risultati sempre peggiori: lo testimonia il dato dello *spread*. Qualche piccolo segnale positivo c'è, peraltro, in questi due documenti che siamo oggi chiamati ad analizzare e approvare: c'è un miglioramento rispetto alle previsioni iniziali e al livello di debito che caratterizza la situazione economica del nostro Paese. Abbiamo però l'esigenza fondamentale di ricondurre il debito su un sentiero di sostenibilità sicura e certa e recuperare la crescita in termini di PIL. Qualcosa non ha funzionato: gli investimenti pubblici non hanno funzionato come ci si aspettava e il loro impatto non è per niente significativo. I tagli alla spesa pubblica devono attenzionarci, perché il rischio è quello di uno scadimento sempre maggiore nei servizi. Mi riferisco

la cultura e la ricerca. Serve, in poche parole, un efficientamento della gestione delle risorse, reso ancora più urgente e necessario dalla paventata compressione delle spese.

c'è un invecchiamento della pubblica amministrazione che mal si allinea con l'esigenza di innovazione e cambiamento che la pubblica amministrazione in quanto tale deve avere. Notiamo questo specialmente nel mondo della scuola,

«pensione sì», «pensione no». Non c'è un attaccamento, ma una disaffezione (specialmente nella scuola) molto pericolosa,

Questa fase di votazione sul bilancio e sull'assestamento apre la fase importante della sessione di bilancio vera e propria. Aspettiamo domani le indicazioni del ministro Tria, ministro Tria, il quale rappresenta per noi un'ancora di salvezza, una persona equilibrata e saggia che ci permette di interloquire alla pari a livello europeo. Spero che manderemo sempre lui in giro per l'Europa e non qualcun altro, altrimenti rischiamo di creare situazioni molto pericolose. Questo dato sul rendiconto non è un aspetto - come diceva il relatore sull'assestamento - puramente formale; è un atto che ha un significato anche di tipo politico, perché da qui partono le considerazioni da adottare nell'ambito della politica di bilancio che dobbiamo approvare. Nella relazione della Corte dei conti al rendiconto 2017 viene indicato che c'è la necessità di effettuare scelte molto caute e interventi di politica economica di tipo selettivo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come il relatore ha indicato, il rendiconto per il 2017 e l'assestamento per il 2018, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, rappresentano gli strumenti attraverso i quali il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria al 31 dicembre 2017 del bilancio 2018. La connessione dei due provvedimenti evidenzia con nettezza che con la riforma del bilancio dello Stato, che il Partito Democratico nella precedente legislatura ha accompagnato e, più in generale, della contabilità pubblica iniziata nel 2009 si sono prodotti importanti passi in avanti. Oggi siamo in presenza di una maggiore flessibilità nella allocazione delle risorse pubbliche e siamo in presenza di una maggiore trasparenza nella rendicontazione delle stesse. Incrementare la flessibilità per ricollocare risorse, scegliere tra risorse e programmi, collocare risorse tra azioni diverse, tra spesa corrente e conto capitale ci ha messo nelle condizioni, nella passata legislatura, di salvaguardare un'iniziativa utile per la crescita e, contemporaneamente, di rafforzare la credibilità e la solidità della finanza pubblica.

Più in generale, quando si eliminano zone d'ombra nella gestione delle risorse pubbliche, il rafforzamento della democrazia può aiutarci anche a un'ulteriore relazione con i cittadini. Insomma, sulla riforma del bilancio dello Stato, della quale attendiamo l'ultimo provvedimento, credo si possa dire di poter operare per un costante rafforzamento degli elementi di flessibilità e di trasparenza necessari per rafforzare la credibilità delle istituzioni. Il rendiconto 2017 certifica la solidità dei risultati raggiunti; rende evidente e credibile l'importanza delle riforme realizzate dai Governi a guida PD per sostenere la crescita. I numeri certificano l'inversione di tendenza importante tra il 2008 e il 2013, il 2013 e il 2017. Lo conferma il PIL, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto; lo conferma la riduzione del rapporto *deficit*-PIL; lo conferma la riduzione della pressione fiscale; lo conferma, in maniera altrettanto netta, l'incremento del saldo netto e, nello stesso tempo, lo conferma e altrettanto in maniera ineludibile ed evidente la riduzione del peso del costo del debito sul PIL. Sarò un inguaribile ottimista, ma auspico con tutto il cuore che la maggioranza Lega e MoVimento 5 Stelle e il Governo del cosiddetto cambiamento cambino narrazioni ed escano dalla retorica dell'inutile e insostenibile accusa al passato. Si metta fine alla campagna elettorale e si operi nel consolidamento di questi risultati. Ci si accorga subito che non è con la decrescita - che, a mio avviso, è sempre infelice - e con un assistenzialismo di annunci che si genera ricchezza, futuro, opportunità e diritti per i nostri figli. secondo auspicio è al limite della sostenibilità del mio ottimismo. Le caratteristiche del nostro bilancio non possono sopportare per nessuna ragione un indebolimento della nostra credibilità, del nostro rapporto tra la dimensione europea e la dimensione internazionale. Occorre ridare credibilità alle istituzioni e - lo dico con tutto il cuore - con gli annunci sbagliati la perdono. Si compromette il peso del debito nel rapporto sul PIL, il costo del denaro per pagare il nostro debito. Entrambi si compromettono anche nel rapporto tra il reddito e il debito delle famiglie e tra gli investimenti necessari per favorire occupazione, lavoro e crescita. Annunciare ogni giorno con un Ministro diverso un diverso incremento del rapporto *deficit*/PIL non aiuta la credibilità del nostro Paese. Cresce la sfiducia nelle famiglie e nelle imprese. Si riduce la propensione ai consumi e agli investimenti. Rinviare provvedimenti per l'emergenza, come sta accadendo a Genova, perché mancano le necessarie coperture, non rigenera la fiducia e non sostiene gli investimenti; si lasciano le persone sole e si perde credibilità nel rapporto con il Paese. Utilizzare la vostra macchina del fango, come avete fatto per aggredire ed impaurire dirigenti della pubblica amministrazione, ai quali va il nostro ringraziamento per la competenza e la serietà del loro lavoro, che hanno evidenziato anche in questo rendiconto e in questo assestamento, non aumenta la credibilità delle istituzioni, ma si produce il caos. E, ancora, isolare l'Italia nella dimensione europea con alleanze anomale e sovraniste, che nulla hanno a che vedere con l'identità dell'Europa, ci isola non solo dall'Europa, ma anche dalla dimensione internazionale e non si attraggono così nuovi investimenti per generare lavoro e crescita, opportunità o futuro; è come respingere la possibilità di credere in un futuro migliore. Così come utilizzare la paura per le elezioni, senza tener conto delle azioni concrete per trasformare la paura in speranza, per trasformare e passare dal rancore e dalla rabbia dentro la dimensione comunitaria, non aiuta i giovani ad individuare un futuro migliore; si possono vincere le elezioni, ma non si fa alcuna azione utile per le generazioni e per il futuro dei nostri figli. Affermare, come ha fatto il ministro Di Maio, che con la legge di bilancio si abolisce la povertà non fa sorridere, perché si offende e si umilia prima di tutto la fragilità delle persone più deboli.

Abbiamo ribaltato una tendenza negativa che ci ha portato a consumare il 9,5 per cento del PIL e abbiamo prodotto un incremento del 3,5 per cento del PIL. Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma dobbiamo partire da questo consolidamento, dalla riduzione della pressione fiscale dalla necessità di rimettere al centro del Paese gli investimenti. Attenderemo tabelle e saldi migliori e giudicheremo con nettezza le azioni sbagliate di questo Governo, proprio perché siamo convinti che lo dobbiamo al futuro e all'amore che abbiamo nei confronti del Paese.

dopo quattro mesi di Governo del cambiamento, non vediamo un grande cambiamento nell'assestamento dei conti, ma spostamenti davvero molto esigui e soprattutto non forieri di particolare rinnovamento nel Paese.

abbiamo l'assestamento e dobbiamo pensare cosa fare per il futuro. Qui arriva veramente il cambiamento: come trovare le risorse per mantenere le promesse immense fatte durante la campagna elettorale, soprattutto dal MoVimento 5 Stelle, che ha promesso qualunque cosa e aumenti di risorse dappertutto. Queste promesse, che uno poteva dire

-, sono state poi confermate nel contratto di Governo, firmato proprio al momento della formazione dell'attuale Governo, dove le valutazioni di spesa sono discordanti, ma sicuramente superiori ai 100 miliardi

e, dunque, qui arriva il cambiamento. Ordinariamente, i Governi quando devono trovare dei soldi, purtroppo, devono aumentare le tasse o ridurre le spese,

decine di migliaia di posti di lavoro verranno cancellati. E se potevano essere errate le valutazioni fatte da coloro che scrissero la relazione per il Governo, parlando

Ma l'innovazione arriva nel modo di trovare questi soldi. Come dicevo, ordinariamente o si aumentano le tasse o si riducono le spese. Questa volta c'è un nuovo modo: minacciare i funzionari del Ministero dell'economia! *(Applausi dal

queste minacce sono state autorevolmente proferite dal potente portavoce del Presidente del Consiglio, il signor Rocco Casalino, Casalino, e le abbiamo potuto ascoltare nelle registrazioni. Questo ha un riflesso su alcuni aspetti della Costituzione, perché l'articolo 97 della Costituzione dice che la pubblica amministrazione deve assicurare l'imparzialità della sua conduzione, per cui o si riscontra una parzialità (per cui si fa un'azione disciplinare nei confronti di quel dirigente) oppure non si può costringere un dirigente, che, essendo un tecnico, ha una sua opinione, ad esprimere una diversa opinione. Anche perché, sempre quel fastidioso articolo della Costituzione, dice che alla pubblica amministrazione spetta di assicurare la sostenibilità del debito pubblico. Per cui, se qualcuno al Ministero dell'economia ricorda che c'è questa esigenza sta semplicemente facendo il suo dovere. Se lo fa, invece, in modo infedele e in modo parziale, allora merita un'azione disciplinare, ma non le minacce attraverso la stampa, sia pure con l'accortezza di dire: no, non l'abbiamo detto noi che siamo al Governo, lo ha detto qualcuno dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Cosa non vera e, pertanto, sarebbe pure una menzogna. momento che il Presidente del Consiglio ha avallato questa posizione e altre figure istituzionali hanno addirittura dato la colpa ai giornalisti, i quali avrebbero dovuto riferire le cose in modo disciplinatamente attinente a quanto detto dal portavoce della Presidenza del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ma la preoccupazione maggiore è dal punto di vista economico. Se espresse in campagna elettorale (si diceva: sappiamo dove prendere i soldi. Noi abbiamo studiato, abbiamo fior di scienziati, di economisti e di professori che hanno studiato tutto. Sappiamo dove prendere i soldi), poi il modo di trovare i soldi è quello delle minacce trasversali,

i litigi all'interno della compagine governativa, e anche al di fuori, hanno fatto sì che fino ad oggi si sia già consolidata una maggiore spesa per interessi (consolidata sulla base delle cifre delle aste della Banca d'Italia) pari a 2,6 miliardi di euro di maggiori interessi che dovranno essere pagati sui titoli già emessi, che hanno una loro scadenza, per cui già c'è stata una differenza di 2,6 miliardi, a contare nel modo più

Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, è con onore ed emozione che oggi debutto col mio primo intervento in quest'Aula. Intervento che ricade all'interno di una cornice finanziaria, tema assai delicato e al contempo farraginoso. Ebbene, è un dato di fatto che abbiamo ereditato un'Italia fragile. Emblematico è il caso in cui versa il sistema viario, compreso quello delle nostre isole - come non pensare alla mia Sicilia - come ha rivelato il caso del ponte Morandi. Ciò impone a questo nuovo Governo delle priorità di carattere finanziario, perché in qualche modo si dovrà pur far fronte

Basta riflettere sull'incremento delle cifre inerenti il livello della disoccupazione e sulla percentuale quasi al 70 della pressione fiscale, per non parlare dell'aumento vertiginoso dei tanti giovani che lasciano la nostra Italia. Si tratta di risorse che perdiamo e di capitale umano che se ne va. Questo è quello che abbiamo ereditato, ereditato, il risultato a cui hanno portato finora tutte le maximanovre finanziarie che avrebbero dovuto rilanciare l'Italia. Dunque, è finito per noi il tempo di giocare con i numeri, quei numeri che hanno mistificato la realtà, perlopiù ingannando i contribuenti, che comunque sono stati sottoposti a un'imposizione fiscale notevole. Penso a quelle politiche di *austerity* che hanno colpito soprattutto il ceto medio, imposte anche dall'Unione europea. Inoltre, i Governi precedenti non hanno saputo rappresentare in modo adeguato gli interessi nazionali in ambito comunitario. È indispensabile una profonda riflessione sulla modalità seguita per i prossimi eletti alle elezioni L'azione politica del nostro Governo vuole finalmente dare volto ai dati numerici e recuperare la dignità dei cittadini, ma prima di ogni cosa vuole conoscere i numeri in modo analitico. Certo, l'idea nobile dell'Unione europea è stata in parte tradita ciò ha creato disaffezione dei cittadini non solo in Italia, ma anche in molti altri Stati europei. Tuttavia, sarebbe ingiusto affermare che l'Unione europea non abbia portato anche dei benefici dal punto di vista culturale e della mobilità dei cittadini all'interno dello spazio Schengen. Ciò ha meritato sicuramente i sacrifici che abbiamo sostenuto. Ma adesso basta, è venuto il tempo di prendere atto della situazione e intraprendere un circuito virtuoso delle effettive risorse di cui disponiamo per il benessere della collettività, nostra unica e sana ambizione. Al contempo, è giunto il momento di rilanciare una nuova idea di Europa, improntata sui principi di solidarietà e condivisione dei suoi originari principi costitutivi. *(Applausi

è faticoso provare ad articolare un ragionamento sul rendiconto e sull'assestamento di fronte al prolungarsi di un lungo messaggio di propaganda elettorale che coinvolge, ancora nelle ultime ore, gli esponenti del nostro Governo. Si molto spesso, segnano la non conoscenza dei numeri e delle situazioni che abbiamo di fronte e che ci mettono un po' di preoccupazione, come ieri sera, per esempio, quando il Vice *Premier*, nel salotto per eccellenza di Bruno Vespa, ha affermato che i Governi uscenti hanno lasciato macerie nel Paese. Nel fare quest'affermazione, Di Maio

avrebbero dovuto ammettere che il documento che oggi essi stessi approveranno racconta un lavoro svolto negli ultimi anni e consegna a chi oggi è chiamato al governo del Paese condizioni di partenza fondamentali ben diverse e più favorevoli di quelle del 2013. Proprio per superare la logica della propaganda, volendo restare al merito, desidero allora subito chiarire che il rendiconto del 2017 tira la linea su quello che è stato l'ultimo triennio dal 2014 al 2017 e fornisce in modo plastico il *trend* dei tre anni precedenti di finanza pubblica, esprimendo tutti gli effetti degli interventi posti in essere, compresa la riforma del bilancio dello Stato; una riforma che ha funzionato e che oggi ci consegna maggiore flessibilità funzionale, ma anche molta più trasparenza nell'esposizione dei documenti di finanza pubblica, quindi di fatto mette in crisi quella propaganda continua ad opera della nuova maggioranza perché sbugiarda punto per punto tutta una serie di *fake news* che continuano furbescamente a distrarre l'attenzione dalle inconcludenze del Governo. Inizio col primo dato: la pressione fiscale. Non è necessario uscire da quest'Aula se l'obiettivo è istigare il primo cittadino arrabbiato e provocatoriamente chiedergli se percepisce che la pressione fiscale degli ultimi anni sia aumentata o no: la risposta "di pancia" la sentiamo anche qui, dentro quest'Aula, dai banchi della maggioranza. Qualcuno, infatti, anche qui dentro, spesso senza nemmeno aver letto, continua ad urlare che la pressione fiscale è aumentata, che è esplosa; lo urla con l'obiettivo di dare in pasto strumentalmente all'antipolitica un boccone ghiotto. Ebbene voi dite

La pressione fiscale, infatti, dal 2014 al 2017 è diminuita dell'1 per cento, nonostante le misure redistributive attuate (vedi gli 80 euro) e che molti di voi non hanno condiviso, men che meno derogato in questo avvio di nuova legislatura. Direte che è poco, che bisogna fare di più; sono d'accordo con voi, ma è ben altra cosa dal dire che la pressione fiscale è aumentata. A maggior ragione non è onesto dire che in Italia, causa dei Governi uscenti, si pagano molte più tasse di prima. Forse sarebbe più onesto affermare il contrario, ma capisco che è chiedervi troppo. Un fatto è certo però: a breve sarete chiamati a dare conto di un esercizio difficile, quello del Governo, che non vi farà sconti. Un'altra bufala che la maggioranza ha cavalcato senza onestà intellettuale, e che anche in questo palazzo riecheggia spesso, è quella per cui in Italia con i Governi a guida PD sono aumentati gli sprechi. Ebbene, data l'impossibilità di trovare in bilancio una generica voce «spreco» (e aggiungo che in questi giorni si intravede bene la difficoltà, in particolar modo di qualche grillino, a scovarli anche nelle stanze di via XX Settembre) è bene sapere che la spesa corrente primaria, dove genericamente si annidano i possibili sprechi, oggettivamente sta passando dal 42,6 per cento del PIL nel 2014 al 41,3 del 2017 ed è la prima volta che si registra l'inversione del *trend* dell'andamento di spesa. È bene dirlo e lo ripeto: è la prima volta. Anche in questo caso si potrebbe affermare che bisognava fare di più. Sono d'accordo, ma è palesemente falso affermare il contrario. Forse sarebbe più utile impegnarsi a provare a fare di più, mostrarsi capaci di fare di più. Potrei continuare così sino ad arrivare al vero *totem* della propaganda giallo-verde: il cerbero del debito pubblico. caso, però, i numeri reali, nonostante le grida, parlano chiaro: il *refrain* secondo il quale con i Governi di centrosinistra il debito pubblico (proprio che quello che oggi si sarebbe disposti a gestire senza freni) è esploso è una bugia. All'inizio del 2014 il rapporto debito-PIL era pari al 131,8 per cento; oggi il documento che discutiamo riporta la stessa percentuale: non è diminuito, ma non è nemmeno aumentato, nonostante importanti misure redistributive. Senza alcun dubbio parliamo di una cifra *monstre* in termini assoluti, che tuttavia ha origini ben più antiche del triennio 2014-2017, che non consentono di piegarla alla propaganda elettorale permanente, dicendo che il debito pubblico è andato fuori controllo. Anzi, dico di più: forse tutti dovremmo sapere che il debito in valore assoluto non potrà diminuire fino a che ci sarà anche un solo euro di *deficit*

Se volessimo semmai essere meno pignoli di Eurostat, come credo dovremmo, ovvero non contassimo gli effetti dell'intervento sul settore bancario, potremmo dire che il *deficit* ha toccato quota 1,9 Anche qui, mi ripeto: sono numeri, sono dati certi e come tali vanno considerati, se solo si ha la pazienza di leggerli. Avviandomi a concludere, voglio esporre solo una considerazione sull'assestamento per Intendo riferirmi all'evidente anomalia relativa alle previsioni assestate di una forte flessione del gettito delle imposte indirette: parliamo di circa 6,3 miliardi di euro in meno. una diminuzione che stona ulteriormente con quell'asimmetria che si riscontra invece nell'aumento delle imposte dirette, che segnano un aumento di 2,6 miliardi di euro. Questa variazione - e concludo davvero - assume un contorno ancora più preoccupante alla luce dei dati pubblicati pochi giorni fa dalla Commissione europea, che riferiscono di un'evasione dell'IVA in Italia, nel 2016, per un totale di 36 miliardi di euro, a cui va da sé associare l'intenzione, più volte comunicata, di voler cancellare lo *split payment*. In questo senso lascio suonare qui, in questa sede, un campanello d'allarme preoccupante, su cui concentrare attenzione e competenza, perché in ogni caso il nostro auspicio, per il bene del Paese, è che possa essere presto contraddetto dall'attuale maggioranza.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, i disegni di legge con i quali si approvano il rendiconto per l'anno 2017 e l'assestamento per l'anno 2018, danno occasione all'Assemblea di esaminare i principali numeri della finanza pubblica, per capire da dove veniamo e dove possiamo andare. È ovvio che sarà il Governo attuale che ci dirà quale strada intende intraprendere, dapprima con la Nota di aggiornamento imminente - ad ore, come si dice - e poi, tra qualche settimana, con il disegno di legge di bilancio per il 2019. I numeri che verranno scritti si dovranno basare proprio sul bilancio esistente, che si può modificare, ma che non si può stravolgere perché è molto ingessato, almeno non con una sola manovra di bilancio.

I principali indicatori sono quelli relativi all'indebitamento netto, che pur diminuendo dal 3 al 2,3 per cento del prodotto interno lordo e scendendo anche in termini reali fotografa quattro manovre in *deficit*, per una cifra complessiva di 172 miliardi Nel contempo, la crescita del PIL è stata di 108 miliardi di euro. Un altro dato da considerare è quello della drastica riduzione degli oneri sul debito, già citati dal collega Ferro, che ha visto scendere da 74 a 65 miliardi di euro gli interessi passivi. L'effetto cumulato è di 38 miliardi di euro di minor onere del nostro debito pubblico. Se vogliamo essere generosi, possiamo dire quindi che il *bonus* di 80 euro, che è costato 6,5 miliardi di euro nel 2014 e 10 miliardi di ai poco più di 10 milioni di italiani che ne beneficiano glielo ha pagato Mario Draghi. Nonostante la disponibilità di tali ingenti risorse, derivanti appunto dal ricorso al debito e dai minori oneri per gli interessi, l'Italia durante gli ultimi quattro anni ha registrato una crescita limitata, al di sotto della media europea. Il nostro prodotto interno lordo nominale ha raggiunto i 1.717 miliardi di euro, uno dei più alti in Europa e al mondo; ma, nonostante questo, la crescita del prodotto interno lordo, trainata da un ciclo internazionale favorevole e da diverse e convergenti variabili esogene, è stata zavorrata dai problemi che ci portiamo dietro da molti anni. È evidente che la crescita economica sia conseguenza diretta della fiducia delle imprese che investono e dei cittadini che aumentano i propri acquisti. È mancata la fiducia, perché sono mancate quelle riforme auspicate da anni e perché si è cercato un improduttivo scontro politico al posto del dialogo. Insomma, se quei soldi presi in prestito dagli investitori stranieri e italiani fossero stati spesi bene, avremmo dovuto almeno avere i numeri della crescita pari a quelli delle risorse impegnate ricorrendo al *deficit*. Così non è stato; non lo è stato nell'ultimo anno, ma nemmeno negli anni precedenti. Così non è stato, riuscendo perfino a sconfessare il cosiddetto moltiplicatore keynesiano. John Maynard Keynes fece un moltiplicatore rispetto alla spesa, vero collega Bonfrisco? Un'ulteriore conferma viene da uno studio empirico, che abbiamo letto anche sugli organi di stampa, circa i 10 milioni di italiani che hanno percepito gli 80 euro, i quali purtroppo non sono ritornati tutti tutti sul mercato dei consumi. Era altrettanto una misura iniqua, perché dava qualcosa a chi già aveva un reddito, mentre non dava nulla ai redditi più bassi o a chi addirittura un reddito non lo aveva. Quella misura mostra un principio di iniquità a chi pensa di mettere sul piatto dell'equità sociale il reddito di cittadinanza, che sarebbe allo stesso modo una misura arbitraria. Prima di tutto sarebbero somme tolte allo sviluppo del Paese, cioè alla creazione di nuovi posti di lavoro, quindi a redditi veri e non di presunta cittadinanza. (vorrei ricordare che noi non siamo contrari all'azione di assistenza a chi ha bisogno). Se realizzate in *deficit*, tali somme sarebbero poi gravate dall'ulteriore onere che pesa sulle somme ricavate dal ricorso al mercato. Parlando di spesa pubblica, va poi detto che anche i consumi intermedi crescono in termini reali e in percentuale più dell'inflazione, assestandosi al 13,3 per cento della spesa corrente al netto degli interessi. Si tratta di una voce importante e ancora molto grigia del bilancio pubblico, perché raggruppa tutto Va evidenziato che purtroppo la centralizzazione degli acquisti non è partita in questo Paese; continuiamo ad annunciarla e speriamo La revisione della spesa allora va realizzata una volta per tutte e noi ci auguriamo che il Governo, ancorché siamo all'opposizione, riesca a realizzarla. Vanno tolti tutti quei vincoli burocratici che impediscono di spendere. Ad esempio per le zone che possono accedere ai fondi

nel recuperare risorse che spesso sono già in bilancio, bisogna fare scelte coraggiose, che indirizzano la spesa non a un consenso immediato, ma a una visione di lungo periodo. In questo desidereremmo vedere quello che non abbiamo visto in questi anni e che non registrano i documenti al nostro esame. Vorremmo essere partecipi di una crescita della spesa pubblica indirizzata all'innovazione e alla ricerca; vorremmo vedere una spesa che passa dalla spesa corrente agli investimenti. A questo punto, uno 0,2 di rapporto *deficit*-PIL può anche diventare molto utile e non irrilevante, in un circuito in cui lo Stato, in accordo con le imprese, si faccia promotore dei processi innovativi. Sapere che in Italia nei prossimi cinque anni mancheranno quasi 300.000 figure professionali specializzate dovrebbe indurre un Governo che guardi al futuro a investire nella loro formazione. Non possiamo permettere che le imprese italiane si trovino prive delle risorse di cui hanno più bisogno, il capitale umano; non possiamo privare gli italiani di tutto ciò. Proprio i numeri del bilancio dello Stato di questi anni dovrebbero indurci a un'inversione di tendenza che pensi concretamente al bene dei cittadini. Quindi, come dice il relatore del rendiconto, non è solo un dato numerico: è la base di analisi per l'attuazione delle politiche pubbliche. Serve una riflessione; abbiamo un Paese ingessato dalle norme dello Stato, dal sistema dello Stato. Serve flessibilità nel riallocare le risorse. Il bilancio dello Stato è lo strumento di finanza pubblica che deve servire ai Governi - e naturalmente a questo Parlamento - come integrazione e surroga di ciò che il sistema non raggiunge.

era l'occasione per mettere mano, da parte del nuovo Governo, al bilancio di previsione del Governo Gentiloni Silveri. Di fatto, non abbiamo visto niente. Vorrei ricordare al nuovo Governo che è entrato in funzione nel mese di giugno, ma da giugno a dicembre ci sono sei mesi e in questo Paese in sei mesi ci sono stati 900 miliardi di euro di

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, graditi ospiti (la nostra generazione *Millennials*), oggi esaminiamo il rendiconto generale dello Stato per il 2017 e l'assestamento del bilancio per il 2018. Il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato» è il dispositivo attraverso cui l'Esecutivo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, realizza l'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 stabilisce che, in allegato al rendiconto, siano illustrate le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura e contenuti ambientali, definite come le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Stiamo parlando dell'ecorendiconto. Le risorse finanziarie destinate dallo Stato alla spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali ammontano nel 2017 a circa 4,7 miliardi di euro, pari, quindi, allo 0,7 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Ma, attenzione: i pagamenti effettivamente realizzati nell'anno sono pari allo 0,5 per cento della spesa primaria complessiva: solo a 2,6 miliardi di euro. Per tutelare il nostro ecosistema, per difendere l'aria che respiriamo, la nostra acqua, la terra, le risorse energetiche e la nostra salute ci si è accontentati di una capacità di spesa pari al 55,4 per cento del totale realmente finanziato. Andiamo nel particolare: per la protezione del suolo e delle acque di superficie e del sottosuolo sono stati effettuati pagamenti per 740 milioni di euro: solo il 28 per cento del totale delle spese realizzate. Per la difesa della biodiversità e del paesaggio ci si è fermati a 411 milioni di euro: solo il 19,9 per cento. Per la gestione dei rifiuti, un tema caldo in nome dell'economia circolare che spesso continuiamo anche a a tirar fuori in quest'Aula, nell'intero anno solo pagamenti per 364 milioni di euro: il 14,1 per cento del totale disponibile. Per capitoli di spesa come la protezione dell'aria e del clima - molto importanti - sono stati emessi pagamenti per appena 60 milioni di euro: pochissimo, sebbene il *budget* fosse ben più ampio e la spesa avrebbe potuto superare i 240 milioni di euro. Nel capitolo su protezione e risanamento del suolo, delle acque e del sottosuolo risultano spesi solo 740 milioni di euro; si sarebbero potuti spendere 1,38 miliardi I contributi pubblici alle imprese avrebbero potuto toccare i 700 milioni di euro, tra trasferimenti correnti (21 milioni) e investimenti pro-ambiente (678 milioni); ma alla fine ci si è fermati sotto i 230 milioni di euro. Permettetemi: questa è stata un'*austerity* non richiesta e io mi chiedo il perché: incompetenza? O forse avete abbracciato questa decrescita felice, di cui ogni tanto vi sento parlare? Dite sempre «decrescita felice», ma secondo me non sapete nemmeno di cosa state parlando. Decrescita felice è il titolo di un libro, scritto da un autore italiano, ma la *degrowth* è qualcosa che si studia a livello internazionale, in tutta una serie di grandi grandi situazioni; anche in America si studia la *degrowth*. È praticamente un modello economico alternativo, si studia con un modello dinamico; andate a leggervi tutta la letteratura scientifica a riguardo e, magari, poi ne riparliamo. Nell'esercizio Ministero dell'ambiente si ritroverà a gestire i lucrosi residui, le somme congelate nel 2017, che si è preferito accantonare: insomma, un vero e proprio tesoretto risorse stanziate, contabilizzate e mai utilizzate, per migliorare la vita dei cittadini e dell'ecosistema. Concludo sottolineando la gravità della dinamica degli investimenti pubblici. Tra il 2014 e il 2017 la spesa per investimenti fissi lordi delle pubbliche amministrazioni è scesa di un ulteriore 0,3 per cento sul PIL, attestandosi a un misero 2 Senza investimenti pubblici non può ripartire quel circuito virtuoso di cui ha urgente bisogno la nostra economia, che, in linea con il resto del mondo, con le *best practice* dei Paesi dell'Unione europea, deve virare verso un'economia sostenibile, *green* e circolare. Gli investimenti pubblici sono un volano, non solo per la domanda nel breve periodo, ma anche per la capacità produttiva potenziale e la competitività delle nostre piccole e medie imprese nel mercato internazionale. Ha ragione il Ministro, quando afferma che oltre 100 miliardi di euro di investimenti sono già scontati nel *deficit* tendenziale, ma non sono stati spesi. La politica del cambiamento è la politica dal volto umano, che metterà fine a una politica disattenta e di austerità, che non ha tutelato le imprese, ha posto poca attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e non si è spesa per migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, dico subito che il Gruppo di LeU si asterrà sia sull'assestamento che sul rendiconto. Solo una piccola notazione: sull'assestamento ci sono variazioni - come già diversi colleghi hanno sottolineato - del tutto marginali. Diciamo che il cambiamento proprio non si vede. Detto questo, per quello che riguarda il rendiconto, forse esso meriterebbe una considerazione diversa, meno burocratica, e probabilmente dovrebbe servire alla maggioranza e al Governo anche in vista della prossima Nota di aggiornamento al DEF. Il quadro che emerge, a ben guardare, è più preoccupante rispetto a com'è stato raccontato: c'è un miglioramento dell'indebitamento netto, ma che sostanzialmente è frutto della diminuzione delle spese per interessi. C'è più trasparenza (questo è un dato positivo), ma rimangono zone d'ombra. C'è una crescita, ma è una crescita che rimane nettamente al di sotto della media europea, ma che soprattutto è diseguale e aumenta diseguaglianze evidenti nel nostro Paese. C'è una riduzione della spesa fiscale, ma rimane impressionante l'evasione fiscale. È di qualche giorno fa il dato dei 36 miliardi di evasione sull'IVA, sull'IVA, cui il Governo del cambiamento risponde con l'evocazione di una pace fiscale/condono e certamente va nella direzione opposta rispetto alle necessità.

con pochi anni fa, un ulteriore *gap* rispetto a tutti gli altri Paesi europei. È un problema molto serio sul quale bisognerebbe riflettere e che dovrebbe portare la maggioranza - vedremo la Nota aggiuntiva - a una riflessione e a scelte di priorità.

francamente penso sia un modo di operare molto sbagliato. Credo ci porterà gravi danni. Sugli investimenti si conferma una caduta. Per quanto riguarda la scuola, uno studio ci segnala una riduzione del 16,3 per cento dal 2009 al 2016 di spesa corrente. Il GIMBE, un centro studi tra i più qualificati sulla sanità, ci dice che dal 2015 al 2018 tra tagli e riduzioni c'è un arretramento di 12 miliardi

che avete un contratto nel quale dite che volete tutelare il Sistema sanitario nazionale e l'universalismo.

quali saranno gli investimenti? Come affronteremo il problema di fare un salto di qualità per dare gambe alla sfida della ricerca e dell'innovazione?

mente. Io non l'ho capito. Va bene la retorica sulle piccole e medie imprese, ma noi abbiamo in manifattura ormai un 40 per cento di imprese che non sono in grado di stare nel mercato. Il mercato interno non tira, non ha la capacità di dare spazio a queste imprese. Che si fa?

di intervenire a «Porta a Porta» o su Facebook, ma con delle norme per ristabilire le cose giuste che vanno ristabilite. Questo è il problema. la nostra discussione è sulla pelle del Paese. anche per questo ci siamo astenuti essendo un fatto sostanzialmente tecnico - quale saranno nella legge di bilancio di bilancio le scelte fondamentali: se non saranno sul rilancio degli investimenti e della spesa pubblica, allora ci sarà poco da fare. Devo poi dire una cosa anche sugli investimenti. Non c'è dubbio che anche le risorse messe sugli investimenti non stanno dando un esito positivo. Dobbiamo chiedercene

necessario uscire dall'equivoco che approvare un rendiconto o un assestamento sia un fatto tecnico. Se si trattasse solo di un fatto tecnico, potremmo rapidamente decidere che forse non c'è nemmeno bisogno di votare il rendiconto, basta pubblicarlo e mandarlo al Parlamento come presa d'atto. In realtà chi approva un rendiconto si assume anche la responsabilità di quello che il documento riferisce e racconta e delle politiche economiche e di bilancio che sono ad esso

lavora anche per dare una vernice di presentabilità ai numeri quando essi rischiano di essere impietosi. A maggior ragione tale ragionamento vale per l'assestamento. Voglio dire, a beneficio soprattutto dei colleghi della maggioranza, che lo approveranno, che un assestamento non è un semplice aggiustamento di conti in corso d'opera che deriva dal fatto che, siccome abbiamo accertato che al 31 dicembre le entrate e le uscite sono quelle, c'è magari una piccola differenza di un miliardo o di mezzo miliardo di euro del bilancio dello Stato, e si tratta semplicemente di riallocare il bilancio di previsione rispetto a quello che abbiamo assestato con il rendiconto.

chi governa verifica lo stato di attuazione dei programmi e delle spese, decidendo se nel corso dell'anno ci sia bisogno di accelerare verso una direttrice, correggere

di previsione. È curioso che invece, quando si assiste ad un nuovo Governo che si presenta come un «Governo del cambiamento» (di cui fa parte un partito che annunciava di volere aprire con l'apriscatole la scatoletta rappresentata dal Parlamento), l'assestamento passi con tre emendamenti. Uno - udite, udite - di mezzo milione di euro; una cifra

per spostarli dalla tutela del paesaggio verso il FUS, sul capitolo dello spettacolo dal vivo. Il terzo emendamento - pensate un po' - è il cambio di denominazione di una tabella. Se questo è tutto il coraggio che avete, oggi il MoVimento 5 Stelle e la Lega approveranno il bilancio di Gentiloni Silveri e Padoan, perché quest'ultimi non avrebbero potuto portare in Aula un assestamento diverso da questo.

Non c'è un solo intervento di cambiamento. Non è mostrato in questo assestamento di bilancio quel minimo coraggio per dire che almeno su una questione, sulla quale abbiamo le idee chiare e su cui

dal Servizio studi, affermando che il bilancio ha assestato più o meno questo e più o meno quello; sono aumentati gli avanzi e sono diminuiti i disavanzi. Insomma, questo leggiamo nelle relazioni tecniche. Politicamente, invece, vorremmo capire dalla maggioranza se il Governo intende davvero cambiare passo. E qui vi annuncio che avete sprecato un decimo di legislatura, perché un assestamento corrisponde a sei mesi di bilancio e una legislatura che dura cinque anni è fatta di dieci semestri. Ebbene, il primo semestre lo avete bruciato così. Voi arriverete al 31 dicembre continuando a spendere i soldi secondo le priorità e gli appostamenti

la prossima settimana o quando sarà pronto il nuovo bilancio, sul quale ci confronteremo, e vedremo che cosa sarete in grado di presentare. positivamente, perché siamo per il bene della Nazione e del popolo italiano. Quindi, facciamo il tifo perché ci sia un Governo capace di rispondere alle esigenze della Nazione e del popolo. speriamo di vedere qualcosa di molto meglio rispetto ai rendiconti che ci sono stati presentati e rispetto ai quali gli interventi trionfalistici del Partito Democratico sono a dir poco surreali. Ma come si fa a vantare la diminuzione del carico fiscale,

politica fiscale. Si scende -udite, udite - al 41,9: quindi, ben 0,8 punti di diminuzione della pressione fiscale. Con questo ritmo ci vorranno ottantasette anni per arrivare a quella pressione tra il 25 e il 30 per cento che un cittadino e un'impresa normale percepiscono come congrua, giusta, equa da pagare e che, quindi, crea una società più civile e più equilibrata.

- come annunciano alcuni ambienti e io spero vengano smentiti - che il primo passo sarà la riduzione di un punto di IRPEF, perché questo lo promettevano pure Gentiloni Silveri e Padoan. Non c'era bisogno di fare

Ma, se leggiamo il complesso del rendiconto di tutta la stagione di Governo del Partito Democratico, dal 2014 al 2017 il rapporto tra debito e PIL 131,8 era e 131,8 è rimasto. cioè, abbiamo avuto quattro anni di Governo passati inutilmente, durante i quali si è affamata la metà del popolo italiano, incrementando la povertà per fasce che non avevano mai conosciuto il problema di arrivare alla fine del mese, mantenendo uguali il rapporto tra debito e PIL, l'indebitamento del Paese

vedrete che cosa succederà con lo *spread*. Questo succede perché ci sono carichi di debito che nessuno ha mai voluto affrontare e che sono la vera priorità del Paese. Per mettere il Paese in sicurezza e al riparo dagli attacchi speculativi,

pronti a difendere il nostro Paese. Lo abbiamo fatto quando, negli anni 2009, 2010 e 2011, la speculazione ha buttato giù un Governo legittimo e qualcuno si fregava le mani e andava in giro per l'Europa tutto contento che questo accadesse.

*(PD)*. Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore del rendiconto e si asterrà sull'assestamento. Prima, durante e dopo la campagna elettorale sono state fatte tante strumentalizzazioni sullo stato dei nostri conti pubblici. L'attuale vice *premier* Di Maio ha parlato più volte di un'Italia sull'orlo del baratro, di un'economia distrutta e di un debito pubblico ormai insostenibile. Anche in questi giorni è tornato alla carica ci ha accusato di essere degli assassini politici e di aver messo il Paese in ginocchio. Che il vice *premier* Di Maio cerchi di recuperare un po' di visibilità nei confronti del vero *Premier* di questo Governo, Matteo Salvini, ci sta, è umanamente comprensibile. *(Applausi dal Il problema è che quelle di Di Maio sono bufale, *fake news*. Basta leggere i dati ISTAT pubblicati cinque giorni fa. Sono dati che ci ricordano che nel 2013, all'inizio della passata legislatura, l'economia italiana era in recessione: diminuiva il PIL, scendevano i consumi, crollavano gli investimenti e l'occupazione e i conti pubblici erano in tensione; il *deficit* sfiorava il 3 per cento e il debito era in aumento, nonostante una pressione fiscale al massimo storico. Quattro anni dopo l'eredità della crisi continua senza dubbio a pesare - non vogliamo sottovalutare la questione sociale e la condizione del Paese, le difficoltà e la sofferenza, che spiegano molto dei risultati elettorali ma l'inversione di tendenza rispetto ai dati del 2013 c'è stata ed è stata netta. Infatti, nel 2017 l'economia è cresciuta per il quarto anno di seguito e sono tornati a crescere non solo il PIL, ma anche i consumi e - ancora di più - gli investimenti e le esportazioni. In questi ultimi anni sono aumentati l'occupazione e le ore lavorate ed è scesa la disoccupazione. Questi dati - intendiamoci - sono anzitutto il frutto del lavoro degli italiani (dei lavoratori e degli imprenditori di questo Paese), della Banca centrale europea e della congiuntura internazionale, ma anche - lasciatemelo dire - di una politica economica che ha tenuto insieme il risanamento dei conti pubblici e il sostegno alla ripresa economica. Non tutto è andato per il verso giusto, perché i dati sulla spesa per investimenti sono negativi. È una tendenza che va invertita quella alla diminuzione degli investimenti pubblici.

che, nel 2017, abbiamo pagato 25 miliardi di tasse in meno rispetto a quanto avremmo pagato con il livello del 2013 *(Applausi

il *deficit* si è ridotto in questo Paese dal 2,9 al 2,4 per cento, che diventa 2 per cento tenendo conto degli interventi straordinari per il risparmio. Certo, c'è stato il calo dei tassi di interesse che ha aiutato molto, ma il grosso di questo risultato, il fatto che il *deficit* si sia ridotto

che si è concentrata non sulle prestazioni sociali, ma sui redditi da lavoro dipendente, sui consumi intermedi, sulle altre voci di spesa corrente. In questi anni, infatti, la spesa complessivamente è diminuita, ma noi abbiamo stanziato più soldi sulla scuola, sulle politiche sociali e abbiamo saputo distinguere la spesa che andava tagliata da quella che andava rafforzata. È questa politica che ci ha permesso di ridurre lo *spread,* che era 270 punti all'inizio della passata legislatura, ed è sceso a 131 punti il giorno prima delle elezioni, permettendoci di negoziare in Europa spazi di flessibilità. Avete vinto le elezioni, siete al Governo. Finalmente nei prossimi giorni dovrete scoprire le carte sulla manovra di bilancio e speriamo - me lo lasci dire, signor Presidente - di non dover attendere come stiamo attendendo il cosiddetto decreto-legge Genova e altri provvedimenti che il Governo ha annunciato, ma che non sono nemmeno arrivati al Quirinale. Da giugno ad oggi, signor Presidente, abbiamo assistito a una sequela di annunci, promesse, parole in libertà: prima il contratto di Governo da 100 miliardi, poi il tira e molla sul *deficit* (sfonderemo il 3 per cento, batteremo i pugni in Europa, ma rispetteremo i vincoli di bilancio e oggi la trincea si è ridotta al 2 per cento). Questo caos - perché di questo si tratta - ha indebolito la credibilità del nostro Paese, non nei confronti dei perfidi mercati finanziari, perché il 70 per cento del debito italiano è nelle mani dei risparmiatori italiani. Sono gli italiani che dovete convincere a sottoscrivere il debito pubblico e li convincerete non con gli annunci, ma se farete una manovra credibile per accelerare la crescita di questo Paese. Per il momento non lo state facendo e questo caos ci costerà caro in maggiori interessi che pagheremo il prossimo anno. Siamo di fronte a un bivio, signor Presidente. L'economia sta rallentando, il sovranismo e il protezionismo a voi cari stanno danneggiando questo Paese, perché l'Italia è un Paese esportatore che ha tutto da perdere dal vento protezionista. Serve una politica economica efficace: il *deficit* non è un feticcio; Keynes ci ha insegnato che è uno strumento di politica economica. Il punto è quanto *deficit* si fa e come lo si usa. Se il *deficit* viene usato in modo intelligente, per fare investimenti pubblici, per finanziare la ricerca, l'istruzione, per dare una mano a chi è veramente in condizioni di bisogno, quel *deficit* innesca un meccanismo virtuoso. Fare *deficit* per diminuire le tasse ai ricchi, fare *deficit* per fare assistenza nei confronti di chi non è in condizione di bisogno è una pessima idea che renderà l'Italia più indebitata e più fragile *(Applausi dal tagliare i soldi alle periferie, tagliare le detrazioni per i mutui e le spese sanitarie - come voi volete fare - non è una manovra del popolo: è una manovra ingiusta. noi avanzeremo proposte alternative attorno ad alcune priorità: le famiglie, i giovani, la lotta alla povertà, il diritto alla casa, gli investimenti. Vi dimostreremo, numeri alla mano, che esiste una strada molto più efficace della vostra per rafforzare la crescita e l'equità sociale, utilizzando al meglio gli spazi di bilancio. Su questo ci confronteremo, signor Presidente, e per questo ci batteremo nella discussione della legge di bilancio.

innanzitutto ricordo l'anomalia di quest'anno. Qualche mese fa abbiamo portato in Assemblea un DEF

sui risultati derivanti da politiche nate magari secondo le migliori intenzioni, ma che non hanno avuto i risultati sperati.

tutte le persone che non hanno avuto, nella loro vita, come famiglie o come imprenditori, i risultati sperati.

soffermerò soltanto su alcuni aspetti, iniziando dalla finanza pubblica. Sul rendiconto si legge che i dati riferiti all'ultimo esercizio, e resi noti dall'ISTAT, attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per il 2017 pari, in valore assoluto, a -39,691 miliardi di euro, corrispondente al 2,3 per cento del PIL, al netto degli interventi sul settore bancario. Quindi, al netto delle disastrose misure salva banche, che hanno avuto un impatto dello 0,4 per cento del PIL, secondo i dati del DEF, il *deficit* per il 2017 si è assestato a -33,184 miliardi che corrisponde all'1,9 per cento del PIL. Quindi, sono dati ben lontani da quelli forniti dal DEF 2018, dove si prevedeva una riduzione del *deficit* all'1,6 per cento del PIL nel 2018. dati che rappresentano l'eredità del PD. La crisi bancaria e le disastrose politiche di salvataggio messe in campo, tramite riforme dal nostro punto di vista sbagliate e certamente portate avanti con troppa fretta, troppa fretta, non hanno certamente portato beneficio al sistema, ma forse hanno agevolato alcuni. Penso - ad esempio - alla riforma del credito cooperativo, che ha accorpato in una *maxiholding* una realtà fatta di piccole e medie banche di credito territoriali, che hanno che hanno rappresentato e rappresentano la vera spina dorsale del settore produttivo italiano e che da sole, durante gli anni della crisi, hanno sostenuto il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, composto - anche se a qualcuno dà fastidio - da piccoli e medi artigiani e da produttori locali Non dimentichiamolo mai. È stata una riforma che ha devastato la nostra rete mutualistica locale e non ha scalfito certamente il sistema dei prestiti alle grandi SpA o alle *mega holding* multinazionali. Tra l'altro, dai dati emersi, al contrario delle previsioni iniziali, le operazioni che hanno coinvolto le banche in difficoltà hanno causato, nel 2017, effetti anche sull'indebitamento netto, per un totale di circa 6,3 miliardi (1,6 miliardi di euro causati dalle operazioni relative al Monte dei Paschi di Siena e circa 4,8 miliardi di euro derivanti dalle operazioni sulle banche venete). Ma anche la Corte dei conti - come ha ricordato qualche collega prima - nel referto al Parlamento sul rendiconto 2017, ha evidenziato delle anomalie e delle incongruenze nella contabilità delle amministrazioni. Ha infatti confermato rilievi critici già emersi negli scorsi esercizi, a causa di diversi fattori: prima di tutto l'esistenza di incongruenze contabili all'interno dello stesso rendiconto delle entrate, essendo stati riportati, aggregati in ordine di importo per titoli, per tipologia e per capitoli, i riaccertamenti e le insussistenze effettuati; in secondo luogo, per la mancata evidenziazione delle riscossioni in conto residui operate nell'esercizio di riferimento, che si trovano invece cumulate con quelle operate in esercizi precedenti e rimaste da versare, incidendo negativamente sulla trasparenza di bilancio. Infine, si è evidenziato, a livello di unità elementare di bilancio, un cospicuo numero di capitoli e articoli per i quali gli accertamenti sono inferiori alle previsioni, sia iniziali che definitive, tanto per la competenza Questa è l'eredità che ci ha lasciato il precedente Governo, alla quale abbiamo cercato di dare un'iniziale ma significativa risposta all'interno del tanto contestato Prima di tutto, sulle banche abbiamo emanato norme di attuazione per il fondo di ristoro finanziario, per rendere effettive le norme messe in atto. A tutela dei risparmiatori, abbiamo accelerato sul tema dei rimborsi, per far sì che i risparmiatori possano avanzare istanza alla Consob per ottenere immediatamente l'erogazione dell'importo liquidato, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro. Un secondo intervento di carattere sistemico riguarda il credito cooperativo: abbiamo cercato di limitare la precedente riforma, per far sì che le piccole realtà mutualistiche locali non finiscano fagocitate dalla capogruppo, per tutelarle dal rischio di trasformarle in una mega SpA, esposta alla possibilità di scalate, anche estere. passiamo ora al tema della pressione fiscale. Nel DEF si leggeva che la pressione fiscale, passando dal 42,7 al 42,5, si è ridotta di 0,2 punti percentuali (l'hanno detto in molti). che riflette l'andamento delle imposte dirette in conto capitale, che sono diminuite in valore assoluto per i minori incassi della *voluntary* *disclosure*, dopo quelli già registrati nel 2016. il collega Misiani ha detto che c'è stata crescita, l'Italia rimane ancora ultima per crescita tra i Paesi fondatori dell'Unione europea e comunque fanalino di coda anche nel blocco dei Paesi orientali, perché rimaniamo in presenza di una pressione fiscale ancora troppo alta, se si vuole davvero rilanciare il Paese. E comunque le imprese italiane sono quelle che versano più soldi nelle casse dello Stato, mentre le famiglie subiscono una pressione fiscale opprimente e non possono usufruire degli stessi servizi dei cittadini di altri Paesi del Nord Europa. Sono state fatte molte illazioni su quello che succederà nei prossimi giorni, a partire dalla Nota di aggiornamento al DEF e poi dalla manovra. Noi abbiamo in mente un altro modo per far ripartire il Paese: certamente cominciare a inserire e ad applicare la *flat tax*. È evidente - ed è stato detto da molti - che non tutto quello che è scritto nel contratto di Governo potrà essere nella prossima legge di stabilità, perché non siamo alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, ma siamo in un Parlamento, di fronte a un Governo che deve presentare dei programmi che possano avere un equilibrio e una fattibilità. Noi siamo consapevoli che questo Paese ha bisogno di ripartire; gli imprenditori e le famiglie ci hanno dato fiducia, il 4 marzo, perché ritengono che noi si sia credibili. Gli imprenditori hanno voglia di ricominciare a rischiare, a riprendere, e con meno tasse. Non è vero che si avvantaggeranno i più ricchi: conosco decine di imprenditori a tutti i livelli pronti a rischiare

perché ci credono, e hanno trovato in questo Governo un motivo per cominciare a sperare. Come dicevo all'inizio, gli elettori hanno sempre ragione: questo sentire si è tramutato in un voto molto semplice, che dà al nuovo Governo il mandato per cercare di cambiare il *trend* di questo Paese e un cartellino rosso e una bocciatura al PD.

del 2017 e sulla manovra di assestamento dei conti pubblici del 2018. Interpretiamo e valutiamo numeri, si potrebbe pensare. E invece vorrei subito sgomberare il campo da questa idea. Nella contabilità di uno Stato, o meglio di una Nazione, che include non solo il concetto di Stato-apparato ma anche il concetto di Stato-comunità, i numeri non sono astrazioni: sono, invece, sintesi di realtà tangibili, fattori che orientano il presente e il futuro di tutti noi cittadini. I dati che oggi esaminiamo ci parlano di spesa pubblica, di investimenti realizzati o mancati, di produzione interna, di lavoro, di pressione fiscale, di servizi resi o non resi ai cittadini. Ci parlano, quindi, di quotidianità, di quanto il Governo precedente - per il rendiconto 2017 - e quello attuale - per l'assestamento 2018 - siano stati capaci di interpretare e soddisfare le aspettative dei cittadini. Appare evidente, dunque, che tali documenti generali riflettono al meglio le premesse e gli effetti dell'azione politica svolta in un determinato periodo di tempo; documenti politici, quindi, non atti tecnici, come qualcuno cerca di farli passare questa sera in questa In tal senso, la nostra sarà una valutazione tutta politica, intendendo con ciò la capacità dei governanti di leggere i bisogni di una comunità, individuare le soluzioni più efficaci e tradurle con coerenza in provvedimenti capaci di incidere positivamente sulla realtà del Paese. ogni modo, segnalare qualche criticità che abbiamo riscontrato come Gruppo politico Forza Italia in merito al rendiconto del 2017. Anzitutto, il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è salito dal 48,2 per

Nel 2017, quindi, il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli, sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. Il risparmio pubblico risulta di meno 12 miliardi di euro, in peggioramento di oltre 3 miliardi rispetto al dato Esso indica che i pagamenti per spesa corrente hanno superato gli incassi registrati sulle entrate correnti. Si riscontra, poi, anche un peggioramento della situazione debitoria a medio-lungo termine per circa 27 miliardi di euro. Si spende troppo, ma soprattutto si spende male, come opportunamente rileva non il sottoscritto, ma la Corte dei conti, critica rispetto all'eccessivo livello di debito del nostro Paese, che ne limita la capacità progettuale di medio e lungo periodo. Da ciò deriva l'esigenza di ricondurre il debito verso la sostenibilità. Noi non siamo favorevoli a politiche di *austerity*, ma siamo per la sostenibilità: il debito deve essere sostenuto, al contrario di quanto sostengono, soprattutto nelle ultime settimane, alcuni importanti e autorevoli membri del Governo. Nulla si è fatto per razionalizzare - ad esempio - le centrali d'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione.

non è stato fatto praticamente nulla in assestamento da parte di questo Governo, anzi. Sono molte le domande che abbiamo posto nel dibattito politico, a partire soprattutto dalla riduzione di trasferimenti ad alcune amministrazioni, soprattutto alle amministrazioni regionali (circa 858 milioni in meno), agli enti di previdenza (1.350 milioni in meno). Come dicevamo, nel corso del dibattito sono state poste numerose questioni anche al Governo relativamente alla riduzione significativa della spesa corrente primaria per trasferimenti e al peggioramento di circa 77 miliardi di euro dell'eccedenza passiva rispetto alla situazione patrimoniale dell'anno precedente. La questione dei tagli alla spesa pubblica ci pare, anche questa, affrontata con superficialità dall'Esecutivo dalla sola prospettiva delle quantità, mentre andrebbe valutata con più attenzione sul versante della qualità dei servizi finali che si vanno a rendere alla collettività; anche questo è evidenziato Questa, cari colleghi, è la fotografia della situazione contabile attuale del nostro Paese. La sostanziale assenza di variazioni in sede di assestamento, laddove invece il Governo in carica avrebbe già potuto varare dei provvedimenti nella direzione di quanto propagandato propagandato in campagna elettorale, è un chiaro indice di *bluff*, perché i numeri raccontano tutta un'altra storia rispetto alle promesse. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ci dicono che mancano le risorse per finanziare tutto quanto è stato promesso e non si è in grado nemmeno di indicare dove andarle a reperire. dell'economia e delle finanze proprio perché non si hanno le risposte. Piuttosto, l'impressione è che sia questo Governo dalla doppia anima a remare contro il buonsenso: si chiedono 30-40 miliardi di tagli, quando la sforbiciata dei tagli alla spesa potrà essere massimo di 3 miliardi; si confonde la manovra finanziaria con un terreno di scontro, a scapito della serietà e della credibilità di un programma unitario e condiviso; si rilasciano dichiarazioni che puntualmente vengono contraddette poche ore dopo, generando caos nei mercati, in cui si bruciano anche i risparmi delle famiglie. Alla prova dei fatti, il peccato originale della propaganda emerge in tutta la sua evidenza: il *gap*, il vuoto fra le promesse e la realizzabilità è incolmabile e bisognerà prima o poi prenderne atto e farsene una ragione. Il Paese ha bisogno di perseguire un programma di sviluppo serio, che incida su fattori strutturali e abbia orizzonti di lungo termine; ha bisogno di uno *shock* positivo, in grado di liberare risorse e indirizzarle nella direzione della crescita, dell'aumento dei consumi, della domanda interna, che dia ossigeno alla produzione e che crei lavoro. Riduzione della pressione fiscale, del costo del lavoro, investimenti in infrastrutture, politiche *ad hoc* per il Sud e per i giovani: sono queste le priorità del Paese, che il programma del centrodestra e soprattutto di Forza Italia aveva posto all'attenzione dell'elettorato; priorità che trovano conferma nei numeri di cui oggi discutiamo, che non lasciano spazio a interventi di assistenzialismo fini a sé stessi. Invece oggi leggiamo addirittura di ipotesi di tagli alle detrazioni per i mutui, spese universitarie e spese mediche, per tentare di racimolare qualche somma che vada a finanziare il reddito di cittadinanza. Purtroppo non ci sembra che il Governo in carica abbia saputo intercettare le reali esigenze del Paese, che chiede sviluppo e non sostegni di sussistenza. L'unico provvedimento importante che abbiamo varato in quest'Aula in questi mesi è stato il cosiddetto decreto dignità, sul quale le previsioni degli analisti e delle associazioni di categoria sono negative e concordi: stimano persino una contrazione di posti di lavoro di circa 120.000 unità. Concludo con un accenno all'ultimo provvedimento, che ha avuto la risonanza mediatica maggiore, soprattutto in questo mese, in questo mese, relativo al ponte Morandi a Genova, su cui ancora oggi non abbiamo le coperture dello Stato. La vicenda è veramente assurda e si commenta da sola. Sono tanti tasselli, dunque, che compongono un quadro preoccupante preoccupante di leggerezza nella gestione della cosa pubblica, di incapacità e di impossibilità di percorrere una strada coerente rispetto a quanto promesso in campagna elettorale. Poiché - piaccia o meno - lo scenario economico nel quale siamo immersi è in rapido peggioramento, come certificato anche nelle ultime settimane dai principali indicatori, il Governo ha il preciso dovere di rendere nota con urgenza al Paese e al mondo la propria strategia. Questi numeri che - come dichiaravo in premessa - non sono simboli o segni grafici, ma espressioni sintetiche della nostra realtà quotidiana, della qualità della vita del comune cittadino come della piccola azienda o della grande impresa, necessitano di essere supportati da un *surplus* di credibilità e affidabilità per reggere il confronto con le aspettative nazionali e internazionali. Il tempo dei desideri vagheggiati è scaduto: se si possiedono strumenti politici per governare con serietà la complessità del reale, è il momento di dimostrarlo. Per questi che - come dicevo innanzi - non sono numeri asettici, sia il rendiconto che l'assestamento di bilancio, ma sono oggi il cuore

il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo rende noto al Parlamento i risultati della gestione di bilancio a metà esercizio, mentre l'assestamento ha lo scopo di aggiornare, sempre a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto. Ci stiamo occupando, quindi, della legge di bilancio per il 2018 che ereditiamo dal precedente Esecutivo e dalla precedente legislatura e che, con ogni evidenza, è il prodotto di visioni politiche ed economiche antitetiche a quelle del MoVimento 5 Stelle. Mai abbiamo condiviso quelle scelte di politica economica, perché non avevano come obiettivo i cittadini, le famiglie e i loro bisogni, né mettevano al centro dell'attenzione e dell'azione politica i giovani, le categorie deboli o svantaggiate, ma obbedivano a formule e assunti che poi si sono rivelati sbagliati, come molti avevano previsto. In questi anni politiche siffatte hanno rovinato letteralmente la vita a tanti italiani - ironia della sorte, mi si consenta di dire amara ironia della sorte - non hanno risolto o avviato a soluzione alcuno dei problemi che affliggono da anni il nostro Paese. Ma tutto questo per noi è il passato. In questi giorni stiamo lavorando per offrire al Paese un reale cambiamento, un radicale cambio di passo. Nelle prossime settimane presenteremo la nostra legge di bilancio, che conterrà misure che riteniamo indispensabili per il Paese e grazie alle quali consentiremo a tanti nostri connazionali, specie a quelli che hanno sofferto in maggior misura in questi anni, la possibilità di una vita migliore, la possibilità di trovare un lavoro dignitoso, la possibilità di sposarsi, di fare figli e di accedere a una sanità e a una scuola di qualità per tutti. Vogliamo offrire loro la voglia di guardare al futuro con fiducia e lo faremo approvando i provvedimenti e le riforme che abbiamo promesso in campagna elettorale e che consentiranno al Paese di crescere in modo sostenibile, di svilupparsi e essere più giusto, più equo e più solidale. In definitiva, approveremo norme nelle materie che costituiscono i punti cardine del contratto di Governo, che questo Gruppo parlamentare sostiene e supporta con convinzione e determinazione. Cambieremo le politiche di ottusa austerità di questi ultimi anni; politiche dissennate che hanno causato un significativo peggioramento delle condizioni di vita di tantissimi cittadini, senza peraltro portare miglioramenti nei conti pubblici, atteso che sono aumentati sia il debito pubblico, sia il rapporto debito-PIL, e, da ultimo, sono peggiorati i dati di cassa, come evidenziati dai *dossier* che sono allegati ai provvedimenti di cui ci stiamo occupando: da questi emerge un peggioramento sia del saldo netto finanziare, sia del ricorso al mercato e, infine, del conto generale del patrimonio. Purtroppo sono numeri: basta leggerli. Cambieremo queste politiche, ma - si badi bene - non abbiamo in programma di sperperare risorse, di fare assistenzialismo di erogare contributi a pioggia. Al contrario, vogliamo eliminare gli sprechi e le enormi spese improduttive. Vogliamo rendere la spesa efficiente e intelligente, capace di avere un impatto positivo e moltiplicatore sull'economia. Tra qualche settimana, quindi, sarà nota la nostra legge di bilancio, che finalmente tornerà a guardare ai bisogni reali dei cittadini e che tratterà i tre temi fondamentali del contratto di Governo: il reddito di cittadinanza, le pensioni e la riduzione della pressione fiscale. Il reddito di cittadinanza ridarà dignità ai tanti italiani che sono senza lavoro e non riescono a trovarlo, perché non c'è offerta o perché non sono formati per professioni richieste in questo momento dal mercato. Questa misura sarà rivolta a coloro che si trovano sotto la soglia di povertà, che purtroppo sono tantissimi nel nostro Paese: circa 9 milioni, di cui 4 milioni in povertà assoluta. Questi numeri sono agghiaccianti e nessun uomo o donna della nostra Repubblica dovrebbe poter accettare come evento fatale e ineludibile. I poveri o quasi poveri che sono aumentati vertiginosamente in questi anni di austerità e i conti falsamente in ordine, certificando in tal modo il fallimento totale di queste politiche che hanno avuto come conseguenza il trasferimento di risorse da chi ha meno a chi ha di più: i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Il reddito di cittadinanza aiuterà tantissimi cittadini a riacquisire dignità e libertà perché, come diceva il presidente Sandro Pertini, «La libertà senza la giustizia sociale non è che è una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame». Diceva ancora il presidente Pertini: «Bisogna che il Governo si adoperi per trovare sorgenti di lavoro, per fare in modo che tutti gli italiani abbiano una occupazione. Questo è quello che deve fare il Governo, questo è quello che deve fare il Parlamento» e noi abbiamo esattamente intenzione di fare quanto diceva il presidente Pertini. Quindi restituiremo dignità e libertà a chi ora non ce l'ha. Il nostro reddito di cittadinanza non sarà una misura *spot*, ma coinvolgerà milioni di italiani, a differenza del reddito di inclusione (REI), istituito dai precedenti Governi. Per ottenerlo occorrerà seguire dei corsi di formazione, lavorare otto ore a settimana per il Comune in cui si risiede e non si potranno rifiutare più di tre proposte di lavoro. Per fare ciò riformeremo anche i centri per l'impiego, che è una misura indispensabile per fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. I centri per l'impiego, del resto, funzionano in tutta Europa, specie nell'Europa del Nord e in quelle Nazioni le risorse e gli addetti impiegati nel settore sono ingentissimi e i risultati lusinghieri sono appunto conseguenti a questi investimenti. Agiremo, inoltre, sulle pensioni: supereremo la legge Fornero istituendo quota 100 e daremo la pensione di cittadinanza. Quindi, le pensioni minime per il singolo cittadino saranno portate a 780 euro. Una parte delle risorse occorrenti le prenderemo tagliando le pensioni d'oro, ossia taglieremo la parte eccedente i 4.500 euro mensili, ma solo a chi percepisce una pensione superiore ai contributi effettivamente versati. Chi, invece, prende una pensione in linea con i contributi versati non sarà ovviamente toccato. Non sarà un esproprio proletario, ma una misura di equità e di giustizia sociale. Non ci fermeremo qui. Vogliamo aiutare le partite IVA, le piccole, micro e medie imprese, che costituiscono l'ossatura produttiva del Paese. Ridurremo la pressione fiscale, che ormai per molti è insostenibile, e spinge molte imprese, artigiani e professionisti a chiudere o, per chi può, a delocalizzare. Inoltre, semplificheranno il sistema fiscale, ma sempre in accordo con i principi sanciti dall'articolo 53 della Costituzione. Gli imprenditori e le partite IVA devono essere liberati dalle scartoffie e dagli inutili adempimenti. Devono poter lavorare e costruire ricchezza per il Paese e devono sapere di dover seguire e applicare poche semplici norme per essere in regola con il fisco e con gli adempimenti richiesti e imposti dalle leggi e dai regolamenti. Però, se sgarreranno o evaderanno il fisco, le pene saranno dure e le sconteranno e - ne siamo certi - questo costituirà un valido deterrente. Qualcuno sostiene che noi del MoVimento 5 Stelle siamo statalisti, non vediamo di buon occhio la libera intrapresa. Niente di più falso e le misure appena elencate lo dimostrano. Cari colleghi e colleghe, quale maggior dimostrazione di amore - mi si consenta il termine - per le imprese del fatto che noi del MoVimento 5 Stelle ogni mese - lo facciamo ogni mese

Grazie a noi nuove imprese sono nate e tanti posti di lavoro sono stati creati. Grazie a noi e ai nostri soldi. Questa è una parte di ciò che faremo nelle prossime settimane. Sono interventi strutturali che hanno come traguardo il medio e il lungo periodo, in modo da dare fiducia e certezza al Paese, ai cittadini, agli operatori economici e agli investitori internazionali. Non faremo commi nella legge di bilancio *ad personam* o "ad aziendam", non daremo mance elettorali: faremo politiche serie, di lungo respiro, come merita il nostro grande Paese. Mi avvio a concludere, signor Presidente. oggi non rispecchiano la nostra visione e i nostri programmi ma, allo stesso tempo, siamo ben consapevoli che la loro mancata approvazione avrebbe gravi ripercussioni sul Paese. sul Paese. Dobbiamo e vogliamo guardare avanti e lavorare nel solco tracciato dal contratto di Governo. *(Commenti dal Gruppo PD).* Concludo ricordando due statisti. Provengo da una terra che ha dato i natali a due grandi uomini delle Istituzioni, a due servitori dello Stato: Aldo Moro e Giuseppe Di Vittorio.

e ho visto foto di Di Vittorio quanto e forse più di voi. Quest'ultimo era un bracciante agricolo, poi sindacalista e parlamentare. Un grande uomo che a causa delle misere condizioni della sua famiglia, non aveva passato molto tempo tra i banchi di scuola, ma che per tutta la vita - prima da sindacalista e e poi qui in Parlamento - si è battuto per i lavoratori, per gli ultimi e per gli indifesi. Era un'altra epoca, un periodo in cui occuparsi dei poveri era un vanto, non come oggi.

Bene, tutto quello che faremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane sarà prendere esempio dai grandi uomini che ho appena citato e faremo tornare i cittadini al centro delle scelte politiche ed economiche.

le comunico che ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, il disegno di legge n. 257, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», è fatto proprio dal Gruppo, avendo le firme necessarie. [DE

annuncio che il disegno di legge n. 603 è stato fatto proprio dal Gruppo. Signor Presidente, colleghi, voglio ricordare che oggi ricorre la Giornata europea delle lingue, celebrata proprio il 26 settembre di ogni anno e istituita dal Consiglio d'Europa per promuovere l'insegnamento delle lingue all'interno dell'Unione. Tra gli obiettivi di questa iniziativa europea, troviamo in particolare la promozione delle ricche diversità linguistiche e culturali dell'Europa, che devono essere preservate e favorite al fine di rafforzare l'integrazione e al contempo valorizzare le lingue minoritarie, ivi comprese quelle meno diffuse. Le lingue regionali e minoritarie, infatti, fanno parte del patrimonio culturale europeo e la loro tutela e promozione contribuisce alla costruzione di una Europa fondata sulla democrazia e sulla diversità culturale. A tal proposito, vorrei ricordare in questa occasione che il primo marzo del 1998 è entrata in vigore la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta dal Consiglio d'Europa e attualmente in vigore, perché ratificata, in 25 Stati membri del Consiglio. L'Italia ha firmato la Carta nel 2000, dopo l'approvazione della legge n. 482 del 1999, che adotta i principi di questo atto internazionale a difesa delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio italiano, ma non ha ancora ratificato la Carta. Proprio per questo ho depositato, insieme ad altri colleghi firmatari, il disegno di legge n. 711, recante «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992», che ripropone, nella sostanza, il testo del disegno di legge di ratifica approvato nella passata legislatura dalle Commissioni riunite 1a e 3a del Senato, il cui *iter* si è arrestato in Aula. Mi auguro che questa proposta possa trovare il consenso di altri colleghi e che questa volta si possa giungere velocemente all'approvazione. Per questo ne sollecito la calendarizzazione, affinché anche in Italia si valorizzi la diversità linguistica come strumento per una migliore comprensione interculturale ed elemento chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro Continente. Vorrei ricordare che in ogni Paese d'Europa ci sono territori fieri delle proprie radici storiche, culturali e di appartenenza a minoranze linguistiche, come quella ladina di cui mi onoro di far parte e di rappresentare. *Develpai de cher*.

un problema che in questi giorni, in particolare la settimana scorsa, ha interessato e sta interessando la zona flegrea attorno a Napoli, con alcuni terremoti di bassa magnitudo, che però si sono verificati nell'area urbana di Pozzuoli, tra la Solfatara e Agnano. Hanno destato una grande preoccupazione perché sono connessi al bradisismo, fenomeno che ha interessato l'area in maniera molto consistente tra il 1983 e il 1985, causando una forte crisi economica in tutta l'area, che si basa essenzialmente sull'economia del turismo e

La nuova zona rossa per i Campi Flegrei comprende, come quella già individuata nel piano del 2001, i territori esposti potenzialmente all'invasione dei flussi piroclastici distruttivi. Che vuol dire? che, in caso di esplosione vulcanica, come si è verificato anche in altro periodo storico, gran parte dei cittadini avrebbero poche possibilità di sopravvivere, per cui la popolazione deve essere evacuata prima dell'evento, dotando la zona rossa di nuove e idonee vie radiali che consentano una facile evacuazione. Significa pure che non si può incrementare il numero dei cittadini esposti al rischio vulcanico, per cui non si possono costruire nuove residenze per ospitare in maniera fissa nuovi cittadini. In una parte del Comune di Pozzuoli, di circa venti chilometri quadrati, si verifica pure periodicamente il fenomeno bradisismico, che causa deformazioni anomale del suolo danneggiando i manufatti che non che non sono stati resi idonei a resistere alle sollecitazioni, che non sono solo quelle sismiche, come già evidenziato nel 1984. Finora non è stata emanata alcuna norma dalle istituzioni competenti che regolamenti l'attività antropica nella zona ad alto rischio vulcanico flegreo. di una zona densamente abitata e credo che ci voglia una disposizione delle istituzioni locali e anche statali che vieti drasticamente la possibilità di realizzare nuovi insediamenti. Concludo evidenziando che questa situazione grave si sta determinando in un momento di crisi dei vertici dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, struttura di grandissima importanza, dotata di ricercatori di altissimo livello che hanno bisogno di una guida trasparente, al servizio di tutti i cittadini. Credo che dobbiamo farci carico della sicurezza di tutti i cittadini. *(Applausi dal

in quest'Aula, vi avevo messo a conoscenza della situazione e del grave pericolo a cui erano stati sottoposti la popolazione e gli operatori civili e militari coinvolti nell'emergenza. Durante il mio intervento avevo sollecitato analisi approfondite sui campioni dell'aria, del suolo, dell'acqua e vegetali, nonché la massima trasparenza nell'affrontare la cittadinanza.

Nel frattempo, giungono continue segnalazioni da parte degli operatori e dei militari coinvolti il giorno dell'incendio che, in modo assurdo, erano privi degli idonei dispositivi di protezione individuale

Tra l'altro, un militare coinvolto sta subendo un assurdo procedimento disciplinare per aver denunciato la cosa al medico competente, senza seguire, a detta dei suoi superiori, la linea gerarchica. Ci siamo attivati immediatamente per avere ufficialmente dai comandi delle Forze dell'ordine, dai Vigili del fuoco e dei militari il reale numero degli operatori coinvolti. Inoltre, chiederemo ufficialmente all'ARPAM tutte le analisi effettuate in questi giorni,

competenti ad attivarsi immediatamente per affiancare gli organi locali e adottare tutti i provvedimenti necessari, anche drastici, accertando contemporaneamente eventuali responsabilità amministrative, civili e penali. Infine, richiedo la massima trasparenza nei confronti della cittadinanza, fino a questo momento assolutamente carente e insufficiente. È una situazione gravissima. *(Applausi dal Gruppo